*(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 24 aprile ricorre l'anniversario dell'olocausto del popolo armeno, perché fu in questo giorno del lontano 1915 che le autorità ottomane decisero l'arresto dell'intera intellighenzia armena (giornalisti, intellettuali, scrittori, persino parlamentari), per poi proseguire con deportazioni di massa della popolazione ed estenuanti marce della morte nel deserto, senza né cibo né acqua, mentre l'esercito turco massacrava il resto della popolazione civile armena presente in tutto il territorio. Ed è per questi motivi che il 24 aprile di ogni anno, in ogni città, paese o villaggio, gli armeni celebrano il Giorno della memoria con una messa, per accostare il ricordo di questi massacri al sentimento del perdono. Se la memoria è, dunque, anzitutto conoscenza, cerchiamo di fare un piccolo sforzo di memoria storica. La storia come memoria dell'umanità, come processo di eventi che rischiano l'oblio, ma che la storia stessa combatte contro il tempo, contrapponendo alla furia degli anni e del silenzio il ricordo e la memoria delle vicende in transito o di quelle già trascorse: è questo il filo conduttore e la grande lezione che dobbiamo ricavare dagli scenari feroci e sanguinari di genocidi come quelli compiuti ai danni di popolazioni innocenti. «Il grande male»: è con queste parole che gli armeni ricordano la data del loro olocausto, una delle pagine più aberranti e, al tempo stesso, più dimenticate della storia. Che cosa accadde tra il 1915 ed il 1916? Per quale ragione in poco più di 12 mesi un popolo che da più di 2000 anni abitava quella terra venne annientato fino a rischiare di non lasciare alcuna traccia Com'è noto, non fu una strage determinata da eventi naturali o da casualità storiche, bensì l'epilogo di uno sterminio, di un massacro pianificato e posto in essere da un preciso gruppo di potere,

? Com'è noto, non fu una strage determinata da eventi naturali o da casualità storiche, bensì l'epilogo di uno sterminio, di un massacro pianificato e posto in essere da un preciso gruppo di potere, per determinate ragioni storiche, politiche ed ideologiche e, soprattutto, con l'intento ben preciso di eliminare la presenza fisica di una nazione - il popolo armeno - e la rimozione della sua cultura. Gli armeni, come le altre minoranze presenti in territorio turco, vennero chiamati alle armi a causa della guerra in atto, ma subito dopo un decreto del gennaio 1915 ne stabilì il disarmo. I militari armeni vennero costituiti in battaglioni del genio: vennero isolati a gruppi di 100, deportati e massacrati. Di 350.000 soldati armeni, nessuno si salverà. Il Trattato di Sèvres del 1920 che sancì l'esistenza di uno Stato armeno indipendente e di un Kurdistan autonomo sembrò riaccendere una nuova speranza per il futuro; così non fu. Mustafa Kemal riprese in mano il vessillo del nazionalismo turco e continuò nell'opera di eliminazione della popolazione armena, iniziata dai precedenti regimi politici. In seguito all'incendio di Smirne, che può essere considerata l'ultima tappa di questo processo di liquidazione, la comunità internazionale si rese scelleratamente complice di questo genocìdio: la Conferenza di Losanna del 1923 annullò gli accordi firmati a Sèvres, le nozioni di "armeno" e di "Armenia" furono eliminate; fu così avallata la pulizia etnica magistralmente operata dai turchi. Ecco perché, nel ricordare oggi l'olocausto del popolo armeno, forse capiamo meglio cosa significa fare memoria di un evento come questo. Di fronte a quello che fu il primo genocidio del Novecento, un crimine negato e dimenticato, ricordarlo costituisce innanzitutto una necessità morale: non come un fatto trascorso in un passato ormai lontano, ma come un evento che ci interpella in modo forte e ci chiama a una memoria viva e condivisa. viva, perché nutrita dall'ansia di conoscere quello che successe e perché porta con sé un desiderio di scoperta non solo della tragedia di questo popolo ma della sua ricchissima storia e cultura. Memoria condivisa, perché consente a ciascuno di noi di sentirsi chiamato a conoscere e a far sapere, al di là delle appartenenze e delle ideologie, il dramma che si è consumato in quei terribili anni di guerra nei confronti del popolo armeno. In un contesto come quello attuale, nuovamente dilaniato da conflitti internazionali, è una grande testimonianza d'amore, una vera e propria lezione di storia farsi testimoni della tragedia di un popolo,

È volgere lo sguardo non altrove, ma dentro la storia, per farsi portatori di una coscienza civile di condanna senza appello di tragedie umane che non dovranno mai più ripetersi. Perché, signor Presidente, un genocidio senza nessuna condanna include e racchiude sempre in sé un grande pericolo: il rischio cioè di diventare una forte suggestione per nuove atrocità future. *(Applausi).*

quotidianamente non si interessa di genocidi, però ci viene a dire che il silenzio sul genocidio più ricordato da oltre cent'anni equivale ad avere silenzi per i futuri genocidi. Questa è un'opera teatrale, una ridicolizzazione di tutti coloro i quali si battono contro gli stermini ed i crimini contro l'umanità per assicurare alla giustizia chi ancora oggi ammazza i propri cittadini. Tutti gli anni viene chiesto di ricordare qualcosa all'interno delle Aule legislative, in Italia e nel resto del mondo, nonché al Parlamento europeo, senza mai però interpellare

quotidianamente studia questi avvenimenti. Quindi, abbiamo una dichiarazione politicamente ancorata ad una lettura di fatti avvenuti quasi cento anni fa che mai ricorda quanto accaduto negli ultimi 18-20, mesi e cioè che finalmente Turchia e Armenia hanno avviato un trattato bilaterale

dimenticato di ricordare come proprio i soggetti citati (addirittura si è sentito parlare di Kemal Atatürk come uno dei responsabili del definitivo sterminio del popolo armeno) hanno invece deciso, di loro iniziativa, contro tutti gli atteggiamenti rigidi che la Comunità europea ha sempre manifestato nei confronti della Turchia, di aprire un dialogo con l'Armenia. Ammesso, e sicuramente non concesso, che tutto quello che ha detto il senatore Asciutti corrisponda alla verità storica dei fatti, quando ci si erge a paladini della memoria di un genocidio occorre sempre ricordare tutta

Oggi, fortunatamente, tutto ciò non è: esiste una democrazia laica in Turchia, esiste una democrazia, molto fragile, in Armenia, esiste - ahimè - un atteggiamento rigido, come quello cui abbiamo assistito poco fa in quest'Aula, che appartiene ai Governi dei 27 Stati membri dell'Unione europea (forse, quello italiano meno rigido degli altri) che insiste nel contrapporre queste due realtà, che invece dovrebbero essere incluse pienamente nell'Unione europea. *(Applausi dal Gruppo

che la Turchia debba entrare a far parte dell'Unione europea, non meno di quanto credo ne sia convinto il senatore Perduca, ma sono altrettanto convinto che le stragi sono stragi. Si chiamano stragi chiunque le abbia

nuova finestra"). Sono presenti in tribuna gli studenti del Liceo classico statale «Socrate» di Roma. Rivolgo a loro e ai loro insegnanti il saluto del Senato

compie gli anni una nostra grande collega. Ne compie 102, ed è Rita Levi-Montalcini ha speso la sua vita al servizio della scienza, della ricerca, ottenendo il premio Nobel, al servizio del nostro Paese e al servizio anche delle donne dell'Africa.

da parte dei senatori Legnini, Belisario e D'Alia - è stata posta la necessità che la Presidenza del Senato assuma una decisione nuova sul nostro calendario, e ne sono state illustrate le ragioni.

A questo momento, quindi a più di 24 ore dall'inizio di queste ripetute sollecitazioni, la Presidenza del Senato non ha ancora fatto sapere cosa ha deciso riguardo alla richiesta

al raccordo funzionale, quindi anche politico, che deve esistere nel lavoro tra i due rami del Parlamento. Credo anche che ci si stia avviando a non prendere una decisione, quindi a presentare

Nei confronti del maggior Gruppo dell'opposizione - parlo per conto del Gruppo del Partito Democratico - quest'atteggiamento è molto scortese. Rilevo che il presidente Schifani, ormai da molto tempo,

e alle quali soltanto lui personalmente può rispondere. Quindi, devo sottolinearlo, e chiederle di riferire al presidente Schifani che considero questa una scortesia che francamente non ci dovremmo aspettare dalla, seconda carica dello Stato. *(Applausi

i colleghi che il presidente Schifani ha comunicato ora che non ritiene di dover modificare le decisioni che sono state già assunte all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo. Questa è la comunicazione, su cui si possono esprimere valutazioni, ma che è stata fatta.

l'intervento del senatore Zanda. Francamente, più che di scortesia politica parlerei di strappo.

Lo farà solo la Camera, e quindi con disprezzo per quest'Assemblea. Dico anche al presidente Schifani, e ai colleghi tutti, che anche a me piacerebbe prendere dieci giorni di vacanza, ma faccio il parlamentare, e ritengo che abbiamo un compito più importante che andare al mare!

vorrei ancora insistere perché la Presidenza del Senato esamini la possibilità di convocare la Conferenza dei Capigruppo per modificare il calendario... partendo dalla piena condivisione circa le responsabilità dell'errore che, altrimenti, tutti assieme compiremmo. È chiaro che la Conferenza dei Capigruppo si è riunita ed ha assunto all'unanimità che, a mio avviso, non corrisponde alle esigenze che la situazione ci detta e agli interessi del Paese. infatti, che la Conferenza dei Capigruppo e la Presidenza del Senato abbiano deciso circa l'inizio del dibattito sul Documento di economia e finanza il 3 maggio nel presupposto che si potessero determinare due condizioni. La prima era che anche il calendario della Camera assumesse quella data per l'inizio dei lavori dell'Aula sul Documento di economia e finanza; richiamo a questo proposito l'intervento molto equilibrato di ieri del presidente Quagliariello che, esattamente su questo punto, ha richiamato l'esigenza di attendere le decisioni della Camera. La seconda condizione era che fosse possibile per il Governo rinviare di qualche giorno l'invio a Bruxelles del Documento di economia e finanza e del Programma nazionale delle riforme in maniera tale da sulla base di una decisione del Parlamento nazionale, intendendo per Parlamento nazionale, signor Presidente, sia la Camera che il Senato, se è lecito sottolineare questo aspetto, dal momento che, anche se a me non piace, siamo in un sistema bicamerale perfetto. Allora - non è responsabilità di nessuno, meno che mai del Presidente del Senato: vorrei che fosse chiaro questo punto - si è assunta una decisione sulla base di due presupposti che entrambi si sono rivelati non esistenti. La Camera ha ormai deciso sul suo calendario: il 28 aprile l'Assemblea si riunirà per pronunciarsi sul Documento di economia e finanza

conferma nel corso dell'audizione del Ministro dell'economia - è che la data del 30 aprile per la presentazione in Europa del Documento di cui stiamo parlando non sarà non sarà superata da nessun Paese europeo, e meno che mai potrà essere superata dall'Italia. Quindi, signor Presidente, oggi stiamo decidendo,

scompaia nell'assunzione di una decisione, come quella riguardante il Documento di economia e finanza e il Programma nazionale di riforma, assolutamente cruciale per il futuro del Paese. Penso che tutto il Senato non dovrebbe la responsabilità di una decisione di questo tipo e, senza polemizzare con nessuno, meno che mai con il Presidente del Senato, ancora una volta invito quest'ultimo a riconvocare la Conferenza dei Capigruppo per rimeditare su un punto che è indifendibile. Ma cosa andiamo a dire, signor Presidente: che non ci siamo potuti

faccio presente al senatore Zanda che l'impegno del presidente Schifani nel presiedere l'Aula, nel seguire i lavori e nell'organizzare le attività del Senato è irreprensibile ed encomiabile. Pertanto, il nostro Gruppo non condivide le parole del senatore Per quanto riguarda il calendario dei lavori, se ne è discusso in due Conferenze dei Capigruppo (in una era presente la presidente Finocchiaro, in un'altra il presidente Zanda), e quindi il calendario, così come è stato definito, è stato approvato. Capisco le osservazioni fatte, ma abbiamo confermato più volte che ritenevamo valido quel calendario e che anche la tempistica della discussione nazionale, parlamentare e europea sui Documenti richiamati in materia economica nulla lede circa il confronto che proseguirà anche con provvedimenti e misure di varia natura.

Chiedo a tutto il Senato, a partire dai colleghi della maggioranza, se esiste un rilievo su un documento di tal peso all'interno della crisi che viviamo e che offre una prospettiva di discussione che durerà anche in Europa.

Perché il Senato, se questo impegno del Governo verrà rispettato, deve essere tagliato fuori da una discussione di un certo spessore che riguarda il nostro futuro,

Signor Presidente, vorrei assumere la sostanza dell'intervento del presidente Marini, il quale si pone il problema

C'è solo un problema da approfondire: se il termine che è stato fissato ‑ questo, presidente Marini, per quel che ci riguarda, ha anche una valenza politica

Ci ha detto che quel termine non è perentorio ma ordinatorio e che comunque non sarebbero stati i tre giorni ad impedire una discussione e un approfondimento.

quindi un impegno a tutto tondo, affinché entro un determinato termine venisse discussa una proposta di legge già approvata in questo ramo del Parlamento. Io non vorrei che dietro questa decisione - ovviamente, presidente Marini, non mi riferisco a lei: il suo discorso è stato assolutamente limpido - si nasconda invece il tentativo di rimandare nell'altro ramo del Parlamento uno specifico punto all'ordine del giorno, sul quale il nostro Gruppo chiederà l'inversione dell'ordine dei lavori. *(Commenti del senatore Morando).* Di fronte all'assicurazione del Ministro dell'economia

gli estremi, né da un punto di vista istituzionale né tantomeno da un punto di vista politico, di rimettere in discussione le decisioni legittimamente assunte dalla nostra Conferenza dei Capigruppo.

non credo dobbiamo nascondere una polemica con un'altra polemica. Il termine perentorio o meno può avere un significato. C'è un adempimento, c'è una legge che è stata votata quasi all'unanimità dal Parlamento e che disciplina questa procedura: si è fissato un termine che, perentorio o meno, ha un suo rilievo di carattere politico e istituzionale che va rispettato. Mi sia consentito però - e non voglio fare polemica nei confronti del senatore Quagliariello - che la circostanza che il disegno di legge sul testamento biologico non sia stato calendarizzato nei tempi richiesti per esempio dal mio Gruppo alla Camera nasce dal fatto

queste sì, collega Quagliariello, che non hanno senso. Non introduca in questa sede questioni ampiamente discusse alla Camera: lasciamole lì, e cerchiamo qui, invece, di lavorare seriamente, cosa che purtroppo da tre mesi non facciamo.

che il termine del 30 aprile potrà non essere rispettato perché l'Italia avrà diritto a qualche giorno in più. Mi sembra l'ennesima brutta figura: noi italiani

il Governo assume questo impegno? Se dovesse assumerlo, noi rispetteremo le nostre ferie; ma se il Governo non può assumere questo impegno, sarebbe una gravissima scortesia istituzionale quella di escludere il Senato dal dare un contributo su un documento che impegna il Governo dinanzi all'Europa. Perché bisogna negare questo diritto all'Assemblea del Senato? Soltanto perché si è deciso che dobbiamo riaprire

sia alla Camera che al Senato

n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché

il Ministro dello sviluppo economico ha preannunciato la propria presenza ai lavori dell'Assemblea a partire dalle ore 12: propongo quindi, alla luce del dibattito che si è instaurato al termine della seduta pomeridiana di ieri, di accantonare l'intero articolo 5 del decreto-legge fino all'arrivo del ministro Romani e di riprendere dall'illustrazione degli emendamenti che si riferiscono all'articolo 6. Poiché non si fanno

Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 6.300. Per correttezza, devo anche dire che ha ricevuto un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81

i livelli essenziali di assistenza all'interno delle quattro ASL, per evidenti fenomeni di instabilità e di mobilità che si sono creati all'interno del sistema sanitario regionale.

il riequilibrio delle risorse economiche necessarie per stabilizzare i precari e garantire livelli essenziali di assistenza avvenga nell'ambito dei fondi complessivi del bilancio regionale destinati alla sanità. In questo, signor Presidente, siamo confortati anche da una sentenza della Corte costituzionale che ha chiarito in maniera molto precisa che la posizione fa sì che le singole scelte per quanto riguarda le competenze nelle spese e nei capitoli di spesa vadano riservate comunque all'autonomia e alla discrezionalità delle stesse Regioni.

riguarda una mera precisazione di un testo approvato dall'Assemblea del Senato con il disegno di legge di conversione del decreto milleproroghe, riguardante i Comuni del cratere aquilano.

i relatori e il sottosegretario Giorgetti, notoriamente molto competente, di dare conferma che non c'è altra modifica o intervento di natura economica. Sull'emendamento 6.0.5 invece, signor Presidente, in ragione di un errore fatto nel disegno di legge di conversione del decreto, noi abbiamo autorizzato una spesa di due milioni per i Comuni dissestati della Provincia dell'Aquila, sempre avendo come riferimento il cratere.

si parla di Regione Abruzzo e non si parla quindi di Provincia dell'Aquila. Si tratta, pertanto, di sistemare da questo punto di vista l'indicazione geografica in modo che tutto

continuare a lavorare e a svolgere dei servizi fondamentali. Tra il *turnover* e la impossibilità di procedere a nuove assunzioni, tutto sommato questi lavoratori, seppure a tempo determinato, stanno svolgendo un importante ruolo all'interno dell'INPS.

ad una semplice variazione di bilancio interna dell'INPS possiamo garantire il lavoro a questi giovani, sebbene, ripeto, a tempo

in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i subemendamenti 5.800/106, 5.800/107, 5.800/110, 5.800/111, 5.800/112, 5.800/113, 5.800/114,

un diverso calcolo del monte a tempo determinato dei precari per gli enti sanitari della Regione Abruzzo, mentre questa norma crea un diritto alla stabilizzazione per una platea di persone indefinibile.

il principio di attenerci rigorosamente al merito delle norme contenute nel testo del decreto. Qui si dovrebbe fare un'eccezione. Poiché si tratta di un'interpretazione, propongo ai proponenti Lusi e Piccone di trasformare

la base di calcolo per operare la riduzione della spesa per il personale precario delle aziende sanitarie abruzzesi non è, come dice la legislazione vigente, il 2009 ma il 2010. L'innovazione legislativa consiste in questo. Il Ministero dell'economia ha sostenuto e scritto poi in norma che questa variazione legislativa non comporterebbe una maggiore spesa. Non si capisce perché il Governo abbia ritenuto, se non c'è una maggiore spesa, di apportare questa innovazione. Non è noto. Ma poiché il Governo evidentemente non credeva a ciò che sosteneva, ha aggiunto

sono noti ai Ministeri dell'economia e della salute, in ragione delle note difficoltà organizzative, anche relativamente al comparto sanitario, legate all'evento sismico: una

mi sembra abbia disatteso volutamente, per spiegare a chi sta votando il senso di questo articolo e di questo comma

di quelli che normalmente aveva. A seguito del decreto-legge n. 78 del 2010, il riferimento ai precari del 2009 penalizzava la ASL di quel territorio in maniera importante, per cui si è adeguato il parametro al 2010, per dare modo a quella ASL di non essere ulteriormente penalizzata.

bene. Rispetto a questa situazione, credo ci siano tutte le condizioni per affermare che è stato riparato in qualche modo un danno indiretto del terremoto, che aveva costretto la Regione Abruzzo a fare riferimento a parametri assolutamente inusuali. Ripeto, è questo il significato della norma,

la sua motivazione mi sembra quantomeno non adeguata alla risposta. Lei, signor relatore, ha detto che vi siete attenuti al criterio di non modificare,

Vede, relatore, la motivazione che ha dato non sta allora in piedi. Non riesco a capire perché - e adesso mi rivolgo al rappresentante del Governo - là dove si tratta di questioni semplici e facilmente risolvibili

al collega Legnini, ma anche alla maggioranza e all'Aula nel suo insieme. Siamo fortemente convinti che la stabilizzazione dei precari non possa avvenire

ci ritroviamo qualche precario assunto in una pubblica amministrazione, tendiamo a stabilizzarlo, togliendo così di fatto il diritto a chi vuole concorrere, ha studiato e si è preparato, di avere un'opportunità.

a riferire in Aula sull'emendamento 5.800, chiedo una sospensione dei lavori. Si tratta di mezz'ora di sospensione.

abbiamo già presentato, oppure se dobbiamo presentarne altri. Dal momento che non abbiamo avuto tempo, tra le votazioni di questa mattina e la seduta in corso, non mi pare che chiedere mezz'ora di sospensione possa portare alcun pregiudizio ai lavori dell'Aula.

Ci auguriamo che il Governo e la maggioranza si aprano al confronto, almeno su quest'articolo, così com'è stato ripetutamente dichiarato in Commissione, visto che su molti punti è stato detto che in Aula si sarebbe cercato di affrontare alcune questioni, anche delicate.

problema che è stato rilevante subito dopo la crisi finanziaria, che è stato in parte affrontato anche dal Governo con alcuni provvedimenti - ricordo che all'interno la Cassa depositi e prestiti è previsto un fondo che deve appositamente sostenere

le piccole e medie imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, che come è noto paga con tempi estremamente lunghi.

indirizzare la Cassa depositi e prestiti a costruire un veicolo societario, dunque una società per azioni che va sul mercato, che può essere partecipata da investitori privati e che fa l'operazione di smobilizzo e di anticipazione di una parte dei crediti della pubblica amministrazione. Dal momento che la Cassa depositi e prestiti costruisce questo veicolo che va sul mercato, partecipato anche da investitori privati, privati, essa risponde per gli interventi che fa in sede di anticipazione per i debiti della pubblica amministrazione nei confronti della piccola e media impresa soltanto con il suo capitale, esattamente come avviene per l'altra parte dell'attività della Cassa depositi e prestiti, che affronteremo successivamente e che riguarda le prese di partecipazione. Quindi, non c'è nessun problema

ad un'esigenza bruciante del sistema delle piccole e medie imprese italiane, realizzeremmo davvero un intervento che aiuta la crescita e che può dare una risposta concreta Il Governo e i colleghi della maggioranza in Commissione non hanno usato argomentazioni contrarie al nostro emendamento. Hanno semplicemente rilevato l'opportunità di avere una sede di approfondimento, rinviando all'Aula i loro orientamenti. Per noi, quindi, è particolarmente importante conoscere l'orientamento del Governo e dei di relatori di maggioranza su questo punto.

Sottolineo che qui è prevista la presa di partecipazione di controllo perché si tratta dell'unica occasione in cui prevediamo che la società veicolo, che la Cassa depositi e prestiti ha già costituito con la modifica dello statuto intervenuta dieci giorni fa,

con prese di partecipazione di minoranza attraverso il veicolo che noi riteniamo debba andare sul mercato ed essere quotato. Ne chiediamo la quotazione non per uno non per uno sfizio di carattere mercantilista - direbbe Tremonti - ma perché vogliamo che tutta l'attività del veicolo che prende partecipazioni sia improntata a criteri di trasparenza, professionalità e rendicontazione al Parlamento. Questo è il senso complessivo degli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 7. Ci sarà anche un emendamento specifico, che abbiamo aggiunto,

finanziario e che quindi sono in condizione, in tempi certi, di restituire la partecipazione alla Cassa depositi e prestiti, affinché non si determinino situazioni come quelle che si sono verificate in passato, non solo con l'IRI, ma soprattutto con la GEPI. Noi insistiamo molto, anche con gli emendamenti, sul fatto che le prese di partecipazione della Cassa depositi e prestiti siano temporanee

l'Italia è piena di casi in cui gli interventi temporanei si sono trasformati in interventi a tempo indefinito. Siccome nel caso specifico parliamo di risorse

società oggetto di partecipazione e sulla temporaneità dell'intervento, e quindi sui tempi di smobilizzo, diventa requisito fondamentale per la presa di partecipazione, perché si agisce con risorse pubbliche.

Detto strumento della Cassa depositi e prestiti opererà in un territorio di confine tra pubblico e privato. Non vi è dubbio infatti che, nonostante la società sia per azioni e quindi sottoposta al diritto ordinario, essendo però partecipata dalla Cassa depositi e prestiti e dalle fondazioni bancarie, abbia una natura sostanzialmente pubblica. Le società che sono oggetto dell'intervento sono private; allora che questi interventi avvengano per decisione non del Ministro dell'economia (perché altrimenti ci troveremo - come abbiamo detto

*board*, quindi del consiglio di amministrazione di questa società (costituito da soggetti aventi alti requisiti di professionalità, di onorabilità e di competenza), e da una tecnostruttura costituita in questo senso, la quale abbia esattamente gli stessi requisiti in modo che gli interventi siano improntati ad una logica di mercato. Non abbiamo niente in contrario a che ci sia uno strumento che opera in questa direzione, ma alle precise condizioni esplicitate, e cioè che operi con un atteggiamento di mercato.

esattamente quanto è previsto dallo statuto della Cassa depositi e prestiti va molto bene, ci convince ma non è una grande innovazione, presidente Azzollini.

ci sarà una relazione del Ministro dell'economia sul tema energetico, cercherò di spiegare perché l'emendamento in questione influenzi in modo particolare il tema, ancora una volta, ahimè, dell'energia in Italia, soprattutto per il versante del gas. Com'è noto, con la decisione che il Governo ci ha comunicato ieri, l'Italia sarà il Paese dell'Europa che marcerà più a gas di tutti gli altri. Circa l'80 per cento dell'energia elettrica prodotta nel nostro Paese ha come fonte primaria il gas; in Italia si consumano annualmente circa 80 miliardi di metri cubi di gas, e poco meno della metà è dedicato alla produzione di energia elettrica. Questo contesto di riferimento va tenuto presente per valutare appieno le ragioni che ci hanno spinto a proporre ancora una volta il tema della separazione proprietaria della rete del gas rispetto al principale monopolista del gas in Italia- io lo chiamo un elemento di innovazione anche nel campo del gas, già ampiamente sperimentato nel settore dell'energia elettrica. Mi riferisco in particolare alla società Terna,

e l'idea stessa di un operatore indipendente nella trasmissione dell'energia elettrica, abbia prodotto nel mercato grazie alla liberalizzazione del mercato dell'energia in Italia. Si può fare benissimo un confronto tra le efficienze raggiunte nell'energia elettrica e le inefficienze, ahimè, presenti invece sul piano del gas.

SNAM Rete Gas doveva essere liberata dalla proprietà dell'ENI e doveva diventare un soggetto indipendente. Come tutti sappiamo, attraverso una disputa, che si è sviluppata prima in sede europea, successivamente in Italia, questo obiettivo è stato sempre rinviato,

Ovviamente, questa decisione è stata il frutto di un compromesso tra i diversi Paesi dell'Unione: da una parte, coloro i quali - gli inglesi per primi - spingevano per un'effettiva separazione proprietaria, e quindi una indipendenza della rete del gas; dall'altra, Paesi, tra i quali Italia e Francia, che in una certa misura resistevano al realizzarsi di questo obiettivo.

ma questa separazione funzionale, come tutti sappiamo, non sarà il regime definitivo, perché il regime definitivo tra qualche anno sarà la separazione proprietaria. Dico perché non è possibile - e ciò che abbiamo registrato in Italia in questi anni lo dimostra - realizzare una effettiva indipendenza, rispetto agli operatori che utilizzano la rete del gas, che metta tutti sullo stesso piano e che quindi realizzi una reale concorrenza, con il risultato di un effettivo abbattimento dei prezzi. perché c'è la rigidità del tubo in quanto tale, che obbliga ad approvvigionarsi da fonti fisse: l'Africa per un verso, la Russia per un altro, la Norvegia per un altro ancora. è poi tutta quella grande massa di gas prodotta in Paesi che non sono collegati all'Italia con un tubo, che ovviamente prima o poi potrà arrivare se si svilupperà la rete

che sarebbe opportuno cogliere l'occasione del cambiamento degli obiettivi e delle finalità della Cassa depositi e prestiti per assegnare alla stessa un'altra missione,

un regime di investimenti infrastrutturali non più legato alle priorità dell'ENI, che ovviamente investe nelle reti se non conviene di più finanziare l'esplorazione di un pozzo di gas; non sempre questi interessi, infatti, viaggiano nella stessa direzione. Soprattutto si potrebbe consentire ai consumatori, all'industria ed anche a chi usa il gas per produrre energia - che, come noto, in Italia è una componente molto importante - di scegliere liberamente il proprio fornitore, potendo contare su un gestore della rete assolutamente indipendente e terzo.

oggi avviamo questo processo, che comunque sarà inevitabile tra qualche anno, tutto il sistema si metterà in movimento, e soprattutto si darà un grande contributo al processo di liberalizzazione dell'energia, in generale,

provvedimento in esame il Governo intende perseguire obiettivi ambiziosi. Si prevede che la Cassa depositi e prestiti possa acquisire partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale sia in termini di strategicità del settore di operatività che in termini di fatturato e di ricadute per il sistema produttivo del Paese. produttivo del Paese. Questa finalità particolarmente rilevante viene poi affidata ad apprezzamenti occasionali, sviluppati in modo episodico, e senza che ciò comporti la misurazione di una sostenibilità e di una utilità nel quadro delle politiche generali su cui il Paese è impegnato. Per tale motivo, proponiamo l'emendamento 7.9, con cui segnaliamo quanto sia necessario per il nostro Paese definire politiche industriali, costruire processi di definizione strategica delle opzioni fondamentali, rispetto alle quali misurare di volta in volta l'opportunità dell'intervento pubblico nell'economia per tutelare quegli interessi che si intendono salvaguardare con l'articolo 7. La vicenda energetica mette in evidenza esattamente questo deficit di visione strategica, perché non è in discussione l'orientamento che una maggioranza doverosamente è chiamata ad esprimere, ma sono necessari strumenti per misurarne la coerenza e perché le politiche pubbliche possano generare quei benefìci, valorizzando in quel modo le potenzialità presenti nel Paese. Con l'emendamento 7.9 che noi proponiamo offriamo dunque al Governo uno strumento per misurare le proprie scelte in termini di valutazione strategica.

Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti 7.4, 7.6 e 7.9. Intervengo sulla parte dell'articolo 7 che possiamo considerare, in ordine di tempo, come l'ultimo capitolo di una storia troppo lunga. che, a nostro avviso, è bene finisca al più presto: quella di un'Italia che, quando le imprese straniere si propongono di investire i loro capitali su grandi aziende italiane, alza le barricate per impedirlo. impedirlo. Per limitarci all'ultimo decennio, abbiamo visto un primo capitolo rilevante di questa storia quando le barricate sono state organizzate dalla Banca d'Italia del governatore Fazio, con il manipolo dei congiurati guidato da Gianpiero Fiorani, contro l'olandese ABN Amro che intendeva acquisire il controllo di Antonveneta.

circa un miliardo che abbiamo speso per tenere in vita con la respirazione bocca a bocca la vecchia italianissima compagnia La quale peraltro è tuttora tenuta in vita giorno per giorno dai viaggiatori che sulle tratte Roma-Milano o Torino-Roma pagano 300 euro invece degli 80 euro che si pagano sulla rotta Londra-Glasgow: ciò è reso possibile da una deroga

E ora la storia si arricchisce di un nuovo capitolo, quello delle barricate contro la francese Lactalis che intende investire su Parmalat.

non è rivolto soltanto a una politica oggi posta in atto da un Governo di centrodestra su questo terreno. Stiamo parlando, semmai, di una

a cui hanno fatto sponda, negli ultimi decenni, la componente più vecchia e conservatrice di Confindustria, da una parte, e la parte più vecchia e conservatrice del nostro movimento sindacale, dall'altra. rispetto a questo farsi sponda a vicenda tra le parti più conservatrici del nostro sistema che occorre voltare pagina. Il risultato di questa storia

un'ideale graduatoria tra i Paesi europei per capacità di attirare gli investimenti stranieri, di intercettarli nel mercato globale dei capitali,

che si colloca appunto a metà di quella graduatoria - ciò a cui noi rinunciamo è l'equivalente del 3,6 per cento del nostro prodotto interno lordo ogni anno; dunque quasi 60 miliardi che potrebbero entrare in Italia e che invece noi teniamo deliberatamente fuori dal nostro Paese. Per intenderci, vuol dire 29 volte l'entità dell'investimento, pur importantissimo, che FIAT, con il suo amministratore delegato Marchionne, ci propone con il piano "Fabbrica Italia". noi non possiamo esimerci dal chiederci perché questi 29 Marchionne restano fuori dal nostro Paese, che cosa ci induce a chiudere loro sistematicamente le nostre porte. È la stessa domanda che finalmente (il fatto va salutato con grande attenzione e favore) ha cominciato a porsi anche Confindustria, qualche responsabilità in quella storia di chiusura tacita protezionistica. Con la costituzione di un comitato investitori esteri presieduto da Giuseppe Recchi, cominciato a voltar pagina interrogandosi su ciò che va corretto nelle nostre politiche su questo terreno. Le risposte che emergono sono in parte ben conosciute: sono il difetto di efficienza delle nostre amministrazioni pubbliche, in particolare di quella della giustizia, con la conseguenza, tra l'altro, di un eccesso grave di burocrazia che affligge chi opera nel nostro Paese; sono i costi dell'energia e dei servizi alle imprese, nettamente superiori nel nostro Paese rispetto agli altri Paesi d'Europa; e anche qui, in questa pessima *performance* del nostro sistema, difetto di concorrenza che nel corso di questa legislatura è stato aggravato da scelte protezionistiche, scelte corporative come quella che proprio in quest'Aula abbiamo compiuto pochi mesi fa in tema di riforma dell'ordinamento forense. protezionistica anche altri elementi, come un sistema di relazioni industriali che gli osservatori stranieri definiscono vischioso e inconcludente a causa del difetto di regole di democrazia sindacale che consentano di dirimere il contrasto che sovente si determina, com'è fisiologico in un sistema di pluralismo sindacale, tra sindacati diversi ma anche fra gruppi imprenditoriali diversi.

di ciò che si sta compiendo oggi, il messaggio che noi lanciamo agli investitori stranieri: se venite in Italia, venite in un Paese delle sabbie mobili, dove appunto le regole possono essere cambiate in corsa; regole inconoscibili per la disorganicità e la non stabilità nel tempo. Collega Tancredi, non prendiamoci in giro. Non nascondiamoci dietro un dito. Questo e non altro è il senso dell'operazione che stiamo compiendo!

ciò che invece il mercato comune europeo è nato per consentire. Perché impedirlo? Sono per garantire a qualche produttore di latte padano la conservazione di una piccola rendita di posizione che potrebbe essere altrimenti insidiata dai concorrenti. Non venga, signor Ministro, a dirci che questo è necessario per esigenze di ritorsioni nei confronti di analoghe norme protezionistiche che in Francia assistono alcune produzioni considerate "strategiche": perché se dobbiamo ridurci a considerare "strategico" lo yogurt e i latticini, allora allora possiamo dire che l'intera costruzione del Mercato comune europeo è stata un errore e che è meglio metterci una pietra sopra. La realtà è che gli investimenti esteri fanno bene a chi li riceve, portano *management*, *know how*, piani industriali innovativi, domanda di lavoro aggiuntiva. Continuando a chiuderci agli investimenti stranieri condanniamo non soltanto l'Italia a non crescere, ma anche i lavoratori italiani a vedere meno valorizzato il loro lavoro. Presidente, la mia illustrazione si traduce in un invito al relatore ed al Governo a valutare il modo di raccordare l'emendamento presentato dai relatori, in particolare il punto *c)* dell'emendamento stesso, con l'emendamento 7.304 nel testo modificato, con il riferimento cioè alle Commissioni parlamentari. In quel caso è evidente che sarei disponibilissimo a ritirare sia l'emendamento 7.304

che punta a riportare nei binari della legge n. 400 del 1988 le fonti che si adottano infatti, un po' troppo frequentemente in questi ultimi mesi e anni viene adottata la formula del decreto non regolamentare che è un modo di assumere pieni poteri senza dover rendere conto né al Parlamento né al Consiglio di Stato né alla Corte dei conti, sfuggendo ai limiti che la legge n. 400 del 1988 poneva in termini garantistici. Questo, soprattutto quando si tratta di una materia così delicata come l'intervento dello Stato in economia con norme che, quando vengono pensate, potrebbero già essere costruite in modo compiuto perché quando si ipotizzano si pensa già a cosa si vuole ottenere. Vorrei pertanto chiudere con il seguente aneddoto. Quando fu eletto alla Presidenza del Cile Salvador Allende, l'allora ministro degli affari esteri cinese Ciu En-lai (oggi si dice Zhou Enlai, perché è cambiata la grafia), gli disse: vacci piano con il socialismo. Ecco, potremmo dire lo stesso al ministro Tremonti: ci vada piano con il socialismo, soprattutto con i decreti non regolamentari. *(Applausi dal

Lungo il corso della sua storia, la Cassa depositi e prestiti ha accompagnato l'infrastrutturazione del nostro Paese, avvenuta in epoche diverse, prima agli inizi del secolo, poi nel dopoguerra. Ricordo a tutti noi che la nostra rete di infrastrutture dell'agricoltura, ad esempio le reti fognarie dei nostri Comuni, le reti energetiche negli anni successivi e quelle idriche (ancor più importanti e sempre più all'attenzione di noi tutti, per quel bene primario che è l'acqua) furono costruite dalle municipalizzate dei nostri enti locali proprio grazie ai finanziamenti a lungo termine della Cassa depositi e prestiti, per arrivare alle reti più importanti e visibili, quelle che utilizziamo ogni giorno, per esempio le reti autostradali, costruite all'epoca da Comuni e Province e oggetto di concessione dello Stato. La riforma della Cassa depositi e prestiti, voluta dal ministro Tremonti due anni fa, ha segnato un passaggio epocale, non solo per il ruolo che la Cassa attualmente svolge, ma per il nuovo ruolo che questo strumento può assumere nel moderno processo di infrastrutturazione del Paese. Il senatore Agostini prima ha ricordato alcuni passaggi importantissimi, la rete delle telecomunicazioni, sulla quale dobbiamo colmare quel *digital divide* che ancora ci separa dal resto del mondo moderno. Ciò può avvenire se la Cassa depositi e prestiti può svolgere il suo ruolo nel modo

che, di fronte a uno strumento di questa portata e di questa importanza per l'equilibrio economico e sociale del nostro Paese, il Parlamento deve poter continuare a svolgere la sua funzione e accompagnare, attraverso una corretta vigilanza, i processi che la Cassa ha davanti a sé, dove occorre intervenire, oppure investire per sostenere i processi di moderna infrastrutturazione, che fanno i conti con equilibri finanziari sempre più delicati e quindi sempre più importanti, mettendo e rimettendo al centro del dibattito economico

opinione) che il ruolo della Cassa sia sempre più orientato verso le infrastrutture che ancora non ci sono, e che noi dobbiamo invece sapere e poter costruire, piuttosto che andare ad alimentare equilibri finanziari su concessioni già collocate, su vecchie infrastrutture, considerato che il processo di apertura al mercato e di liberalizzazione può tranquillamente assegnare questo ruolo al privato che investe nelle infrastrutture pubbliche, mentre considero importantissimo il ruolo che la Cassa depositi e prestiti può avere per il futuro del nostro Paese. nostro Paese. A questo proposito, il ruolo del Parlamento non può venire meno. Il Parlamento, attraverso una Commissione di vigilanza che elegge all'interno dell'Aula, con una votazione che demanda ai parlamentari eletti il ruolo di vigilanza, può può avere oggi alcune garanzie. Deve averne di ulteriori, secondo me, perché quei poteri e quel ruolo sono ancora stabiliti da un regio decreto del 1913. Se la Cassa depositi e prestiti è lo strumento più efficace e moderno che il nostro Paese mette in campo per l'infrastrutturazione del Paese, è giusto, secondo noi, che

sugli investimenti, le scelte e le decisioni della Cassa depositi e prestiti. Se questa è la strada per la quale si vuole arrivare a congiungere una visione moderna e puntuale del ruolo del Parlamento con il nuovo ruolo della Cassa depositi e prestiti, si faccia pure, e si contempli in un unico testo il ruolo della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti eletta dalla Camera dei deputati e dal Senato, per espletare quella funzione di controllo e vigilanza che non potrà più essere solo *ex post*, ma dovrà essere anche *ex ante*.

questo dibattito si svolge quaranta giorni dopo il disastro che ha colpito il Giappone e l'incidente gravissimo della centrale di Fukushima; giorni che hanno aperto un ampio dibattito a livello mondiale sulla produzione di energia da centrali nucleari, e che il Governo italiano ha utilizzato per dare coerenza alla propria strategia di approvvigionamento energetico. quarant'otto ore dopo l'incidente tutti i Governi europei, compreso quello italiano, sono stati convocati a Bruxelles per approfondire l'emergenza creata dall'incidente di Fukushima ed immaginare soluzioni, anche se fin dall'inizio si è registrata disomogeneità fra i diversi Paesi, pur nella comune esigenza di rafforzamento delle misure per accrescere i livelli di sicurezza e di standardizzazione. Ad oggi abbiamo Paesi come la Germania, che hanno portato già a conseguenze molto avanzate l'esigenza di rivedere la mappa delle proprie centrali, con particolare riguardo a quelle di prima costruzione, e Paesi come la Francia, che spingono sulla revisione ma non chiusura dei propri impianti, per alzarne invece il livello di sicurezza.

Proprio la definizione dei parametri di sicurezza, che dovranno essere condivisi da tutti i Paesi e proposti, com'è intenzione, ai Paesi extraeuropei, è la priorità che le agenzie per la sicurezza dei diversi Paesi devono ora affrontare e risolvere. Soltanto dodici giorni dopo l'incidente, il Consiglio dei ministri del 23 marzo decideva di inserire in un decreto-legge la cosiddetta moratoria, ossia la sospensione dei termini del programma nucleare già definito in precedenza, per dodici mesi. Una riflessione ritenuta opportuna proprio per garantire l'allineamento alle procedure europee prima citate. Negli stessi giorni il Governo ha dato impulso alla creazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, della quale stiamo ora definendo gli aspetti organizzativi, con l'obiettivo di partecipare a pieno titolo al processo di analisi e definizione degli *standard* di sicurezza. Tutto ciò è dimostrato dagli sviluppi del decreto-legge in prima una disposizione con cui è stata prevista la moratoria di un anno rispetto all'attuazione del programma per la realizzazione di impianti nucleari; poi l'emendamento presentato ieri, coerente con la decisione della moratoria, che ne sviluppa le conseguenze. Un serio approfondimento sui profili di sicurezza della produzione di energia da fonte nucleare non può essere vincolato a termini temporali, in ogni caso predefiniti. Occorre predisporre le condizioni perché possa avvenire nel modo più sereno e proficuo. Del decreto legislativo n. 31 del 2010 e del decreto legislativo correttivo n. 41 del 2011 sono mantenute soltanto le disposizioni che riguardano il trattamento dei rifiuti e delle scorie radioattive derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e il *decommissioning* degli impianti pregressi. È evidente, infatti, che si tratta di attività importanti e delicate, che prescindono dalla realizzazione o meno di impianti nucleari e che è necessario svolgere nelle condizioni migliori possibili. Nel frattempo, secondo le peggiori previsioni, la situazione della centrale di Fukushima non si è purtroppo normalizzata, anzi il livello di rischio è salito a quello attribuito all'incidente di Chernobyl. E la situazione è ancora in evoluzione. L'Italia si trova in un Continente che ha già fatto la sua scelta per la produzione di energia nucleare: energia che importiamo e che viene prodotta ai nostri confini. Il nostro percorso di rientro nel programma nucleare, come era stato disegnato, era coerente con quel quadro e con le nostre esigenze energetiche. Ora quel quadro è drammaticamente cambiato, e coerenza vuole che la riflessione tempestivamente aperta nel nostro Paese si tramuti in una strategia di revisione del programma stesso prevedendo: innanzitutto, una partecipazione a pieno titolo alla costruzione europea dei nuovi *standard*; in secondo luogo, una presenza industriale legittimata da una filiera esistente in Italia e che si stava preparando ad un suo rafforzamento; in terzo luogo, uno sforzo scientifico di approfondimento delle soluzioni avanzate per il «nuovo nucleare» europeo. Quindi, una partecipazione a pieno titolo delle nostre istituzioni scientifiche e di ricerca, delle aziende della filiera nucleare, ai nuovi criteri che saranno stabiliti in Europa per le centrali che i singoli Stati, ma in un processo di coordinamento europeo, decideranno di mantenere in funzione. Quindi, il quadro di compatibilità nucleare per l'Italia potrà essere chiaro solo dopo questi passaggi: è questo già un motivo ampiamente sufficiente per rinunciare oggi all'impostazione data nel 2009 e rinviare una decisione così importante al chiarimento complessivo in sede europea. Ecco perché riteniamo che gli stessi cittadini sarebbero stati chiamati a scegliere fra poche settimane fra un programma di fatto superato o una rinuncia definitiva sull'onda dell'emozione, assolutamente legittima dopo l'incidente di Fukushima, senza avere sufficienti elementi di chiarezza. In Europa, inoltre, dobbiamo essere forti di una strategia definita per avere voce in capitolo, non essendo un Paese con impianti nucleari sul nostro territorio. Ricordo che 14 Paesi su 27 non hanno impianti nucleari, ma l'unico grande Paese a non averne è proprio l'Italia. La campagna referendaria, e a maggior ragione un esito abrogativo del *referendum*, avrebbe messo decisamente in secondo piano le nostre posizioni, le richieste, le pressioni con cui vogliamo garantire invece sicurezza al nostro Paese. La sindrome Nimby (*not in my backyard*) non ci deve travolgere. Noi dobbiamo parlare in Europa a pieno titolo perché la sicurezza dei nostri cittadini dipende dalle centrali installate in tutta Europa. Il *referendum*, al contrario, non può abrogare al di fuori dei confini nazionali; non impone parametri di sicurezza, e quindi non dà nessuna garanzia di poter decidere *standard*, parametri, criteri validi per noi ma soprattutto per gli altri. Ora si apre una fase ulteriore che impegna Governo e Parlamento nella scelta di un piano energetico nazionale in grado di garantire i consumi del Paese - previsti in aumento con l'uscita dalla crisi - a costi sempre più sostenibili per le famiglie e per le imprese. L'emendamento 5.800 infatti ridefinisce i contenuti della Strategia energetica nazionale che il Governo è chiamato ad adottare, eliminando peraltro il riferimento alla produzione di energia nucleare, in coerenza con le precedenti disposizioni dell'emendamento medesimo. La Strategia, sulla base degli obiettivi e delle indicazioni fissati dall'Unione europea e dai competenti organismi internazionali, deve rispondere ad alcune esigenze fondamentali, alle quali per lungo tempo non si è prestata l'attenzione necessaria, con conseguenze pesanti dal punto di vista economico. La prima esigenza a cui far fronte è quella relativa alla sicurezza della produzione di energia e alla sostenibilità ambientale; la seconda è quella che fa riferimento all'idoneità dell'approvvigionamento energetico sotto il profilo quantitativo, all'economicità per le famiglie e per le imprese e, al tempo stesso, all'attenuazione delle condizioni di dipendenza dai Paesi esportatori di petrolio e gas. Per raggiungere queste finalità occorre impegnarsi per il potenziamento delle infrastrutture energetiche, per il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo e per la promozione e valorizzazione delle filiere energetiche nazionali. Ed è chiaro che le attività di ricerca interesseranno il settore energetico nel suo complesso e saranno finalizzate a sviluppare tutte le soluzioni che potranno favorire il conseguimento degli obiettivi indicati. È di un disegno complesso, da cui dipendono in misura importante le prospettive di sicurezza e benessere del Paese. Per questo, se da un lato è compito del Governo dimostrarsi in grado di delineare la strategia, dall'altro essa deve essere oggetto di riflessione, di confronto e, auspicabilmente, di condivisione nelle sedi istituzionali più qualificate. L'emendamento 5.800 prevede in proposito che la proposta del Governo sia sottoposta all'esame della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari. Ora l'obiettivo - e non voglio rileggere il comma 8 dell'emendamento, che immagino conosciate bene - è quindi la ridefinizione della strategia energetica nazionale che, nell'alveo di quanto disposto dalla legge e prendendo in considerazione le disposizioni europee, sia in grado di garantire la diversificazione, anche sotto il profilo geografico, dell'approvvigionamento relativo alle fonti tradizionali, la promozione delle energie rinnovabili e l'appropriata considerazione dei risultati a cui porteranno gli approfondimenti di carattere scientifico e tecnico in materia di sicurezza del nucleare.

l'intervento del senatore Rutelli, che aveva detto: ma cos'è questa perplessità in Aula? Cosa significa? Rallegriamoci del fatto che il Governo finalmente ha capito di dover prendere una svolta su una decisione sbagliata.

Però non nascondo che mi rimane la preoccupazione che tutto questo, non dico che sia una truffa, come ha scritto qualcuno oggi sui giornali, ma una mossa molto tattica per evitare il *referendum* che si terrà il 12 giugno. Ieri

I costi per un impianto come quello di Olkiluoto, l'unico reattore di terza generazione, sono aumentati a 4,5 miliardi di euro.

che sono i più grandi produttori di uranio. E le risorse dureranno,

Quanto stiamo spendendo noi per le rinnovabili in Italia? Invece di aumentare gli interventi, cosa ha fatto il nostro Governo? Ha ridotto i contributi per le rinnovabili, mentre tutti, compresi i parlamentari della maggioranza, si erano sforzati, anche in Commissione, di rimarcarne

al quale mi sono permesso, insieme al collega Ferrante, di presentare un'interrogazione. Ma attenzione a questa discussione. Non si tratta solo di energie rinnovabili. Si tratta di compiere tre scelte, di cui la prima è quella del risparmio energetico, la seconda è quella dell'aumento dell'efficienza dell'energia e solo la terza attiene alle rinnovabili. Mi soffermo sull'aspetto del risparmio. Avevo già citato un esempio. La provincia di Bolzano la casa clima ha sviluppato molto di più di un'alternativa: ha sviluppato un marchio ormai europeo, addirittura mondiale, esportabile.

ultimo, spendere una parola di moralità, se in quest'Aula si può ancora fare. Ma questa generazione è talmente egoista da non capire che i nostri figli avranno un pericolo grandissimo grave che penderà

Signor Presidente, signor Ministro, la discussione che stiamo ora affrontando, e che è stata aperta dall'intervento appassionato del collega Peterlini

di una discussione necessaria e propedeutica alle votazioni che faremo oggi e pregherei il Ministro di dedicare attenzione al dibattito. Perché questa

attraverso gli emendamenti presentati e alla luce della svolta determinatasi ieri, dopo la presa di posizione da parte del Governo, dovremmo decidere esattamente che cosa si fa, e mi spiego. È evidente a tutti che, poiché questa decisione interviene in pendenza di un *referendum* abrogativo, abrogativo, la volontà politica e istituzionale del Governo e della maggioranza, sottintendente le sue determinazioni giuridiche,

sostanziale in materia, sarebbe molto difficile per la Corte di Cassazione, chiamata a valutare, una volta che le norme venissero licenziate, dal Senato prima e dalla Camera dei deputati poi, se tali norme siano in grado di

ma ad una sospensione, il risultato sarebbe esattamente quello che si sarebbe registrato nel caso in cui fosse stata votata la norma inizialmente proposta dal Governo, ovvero una sospensione per un anno del programma nucleare. a parere di chiunque conosca la giurisprudenza della Corte di cassazione in questa materia, che nessuna norma di mero differimento della materia avrebbe la capacità di provocare un effetto di soppressione della scadenza referendaria, ragion per cui il *referendum* si terrebbe comunque interverrebbe una decisione, che in ogni caso spetta all'organismo preposto, che è la Corte suprema di cassazione, per giudicare se gli obiettivi dei promotori del *referendum* siano stati conseguiti oppure no. Ebbene, c'è un solo modo per conseguire l'obiettivo, signor Ministro: quello di abrogare le norme, ovvero di ottenere con estrema chiarezza e precisione lo stesso effetto che il *referendum* determinerebbe.

la materia riprodotta dal quesito del *referendum*. Lo dico perché, per usare una battuta comprensibile a tutti, non si può essere, come si diceva un tempo, un po' incinte: o c'è l'abrogazione o la sospensione. Non ci può essere una quasi abrogazione e una sospensione un po' più decisa: o si prevede l'abrogazione,

oppure la si sopprime interamente. Ma a quel punto, signor Presidente, è evidente che toccherà al Parlamento, come è già avvenuto, legiferare su un nuovo programma energetico complessivo, e non certamente ad un decreto governativo di qualunque rango, da sottoporre meramente all'esame delle Commissioni parlamentari.

conseguente agli eventi di Fukushima, ma da un'analisi che l'intero mondo economico, produttivo e scientifico che si occupa dell'energia nucleare ha dovuto avviare dopo la tragedia di Fukushima. Ricordo che, all'indomani dell'incidente alla centrale statunitense di Three Mile Island, gli Stati Uniti d'America fermarono per un quarto di secolo qualunque nuovo programma di installazione di centrali nucleari. È evidente che gli eventi di Fukushima hanno dimostrato - come ha poc'anzi ricordato il collega Peterlini

il raffreddamento delle centrali non è ancora ripartito e le procedure di messa in sicurezza impiegheranno, secondo le autorità giapponesi, ancora tanti mesi, (non si sa quanti) per non parlare del recupero delle condizioni di vivibilità nell'area dei

salta il programma nucleare italiano non solo perché le centrali sono insicure, ma perché l'innalzamento, peraltro in un'area ad elevata sismicità qual è la nostra, requisiti di sicurezza avrebbe un costo incompatibile con le nostre esigenze. Non dimentichiamo che il programma nucleare italiano, destinato a soddisfare il 25 per cento del nostro fabbisogno elettrico,

- fase - per soddisfare quel fabbisogno, e ciò sarebbe totalmente sproporzionato ed insostenibile. Signor Presidente, ciò che è avvenuto negli anni passati è privo di trasparenza, perché il Governo non ha mai detto in

raggiungere i *quorum* su altri *referendum*. Oggi ci occupiamo del nucleare, e su di esso c'è una presa di posizione di un'importanza straordinaria, che ci proietta, signor Presidente e signor Ministro, in una direzione nuova, completamente nuova. Sono d'accordo anche sull'orizzonte europeo. Credo che l'Italia debba proporre una sorta di Comunità europea, come fu alla nascita

di mettere in comune i tubi per la diffusione del gas, ma, soprattutto, dell'autosufficienza energetica dell'Europa e dell'Unione europea. È un grande orizzonte al quale l'Italia arriva con la fortuna di non avere sul groppone 35 miliardi da spendere in un programma vecchio, obsoleto e oggi fallito. Quindi, guardiamo con più speranza futuro e a questa pagina di oggi come un grande appuntamento che segna una svolta per la politica energetica e ambientale nel nostro Paese. Presidente, onorevole Ministro, colleghi, chi non muore si rivede. E si rivede a stretto giro di posta. Voglio subito fare una precisazione per evitare spiacevoli confusioni: è da un anno che l'Italia dei Valori ha costretto il Paese - per Paese intendo la politica e la società nelle sue molteplici e complesse articolazioni a discutere dell'energia nucleare. Noi non avevamo e non abbiamo un approccio ideologico all'energia atomica, ma sappiamo, signor Ministro, che il nucleare sicuro è quello che non c'è. Per questo, il mio partito, da solo, è al servizio del Paese da un anno a questa parte raccogliendo le firme per il *referendum* abrogativo, non tanto e non solo delle norme che consentono - lo dirò più avanti - il ricorso al nucleare, ma per mettere un altro punto esclamativo alle cicliche e dannate conversioni sull'energia mortale nucleare. Un primo punto fermo noi italiani lo avevamo messo nel 1987, ma l'arroganza, la cecità e l'interesse di questo Governo ci avevano portati verso un vicolo chiuso. Oggi siamo lieti che tanti - tanti davvero - siano venuti sulle nostre posizioni e siamo ancora più lieti che il problema della produzione di energia nucleare sia posto all'attenzione dei cittadini italiani con le criticità, le preoccupazioni e le paure che gli italiani hanno. il Governo ha scelto strade diverse e poi, quasi folgorato sulla via di Damasco, dopo un decreto in cui in cui aveva parlato di moratoria nucleare e molteplici apparizioni in quest'Aula (l'ultima è avvenuta il 7 aprile 2011, quindi ben oltre l'11 marzo del 2011), ha sostenuto la indifferibilità e la necessarietà di questa scelta. Il ministro Prestigiacomo lo ha detto ieri; il ministro Gelmini lo ha detto ieri; il ministro Matteoli lo dice oggi: il Governo non ha alcuna intenzione di abbandonare il nucleare. Ha scritto una norma di moratoria in maniera diversa, come adesso dimostrerò. D'altra parte, con i Resoconti parlamentari, con la relazione del Ministro e con l'interpretazione autentica della volontà del Governo, la

del nuovo nucleare europeo, al quale noi partecipiamo, della filiera del nucleare, del rinvio del nucleare. Voi il nucleare non lo volete

il suo intervento, ci troveremmo di fronte - ma con questo Governo, mi consenta, Ministro, non ci meravigliamo - ad una truffa colossale, ad un imbroglio epocale, ad una patacca una patacca monumentale, ad un gioco delle tre carte indegno di un Governo serio. ricordare che al primo comma di questo emendamento 5.800

mio Gruppo - si farà rientrare dalla finestra quel che voi fate uscire dalla porta. Questo non è, perché dobbiamo mettere una parola finale: diversamente, noi andremo al *referendum*. La preoccupazione vera, ministro Romani, per questa soppressione, è non portare il popolo italiano a

la sua politica giudiziaria, per affrancarsi, sempre e comunque, dalla sua posizione di plurimputato. Ecco perché, o il Governo metterà una parola fine determinata, altrimenti, come ha scritto una raffinata penna come quella di Gramellini, se io fossi un nuclearista mi sentirei seccato da questa repentina girata di tacchi che non è stata nemmeno motivata. Anzi, in quest'Aula, e i Resoconti ce lo diranno, il Governo ha detto: «Attendiamo un momento, imbrogliamo il Paese, e poi ritorneremo al nucleare». Per questo, signor Ministro, il Governo, per non fare il *referendum* dia parere favorevole agli emendamenti che l'Italia dei Valori ha presentato che cancellano definitivamente il nucleare. Altrimenti si voti. Quando lo si farà

Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le gravi vicende dei reattori giapponesi impongono una pausa di riflessione sullo sviluppo dell'energia nucleare nel nostro Paese. L'emendamento presentato dal Governo al decreto in discussione è una chiara presa di responsabilità da parte dell'Esecutivo ed accoglie le aspettative dei cittadini in merito ad un'ulteriore riflessione su una problematica che mai come in questi giorni suscita preoccupazione ed incertezza. L'intervento del Governo si allinea con gli orientamenti degli altri Paesi europei che stanno rivedendo le loro politiche energetiche al fine di garantire un più alto livello di sicurezza

un grande piano europeo per le fonti rinnovabili e la ricerca di energie alternative con riferimento ad una analisi economica che tenga conto, oltre che dei costi relativi allo smaltimento e messa in sicurezza delle vecchie centrali, del calcolo del rischio radioattivo, poiché se è vero che i benefici a livello locale sono inconfutabili, le ripercussioni negative generali sono forti. Resta di fatto la necessità di approfondire la tematica relativa alle fonti energetiche rinnovabili, quali fonti di importanza strategica per la protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. La Lega Nord, nel sostenere l'opportunità strategica per il Paese di approfondire lo studio di una politica energetica fondata sul nucleare, ritiene comunque indispensabile sviluppare piani energetici che tengano conto delle fonti rinnovabili anche ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti nell'ambito del mercato interno dell'elettricità, come segnalato in una recente mozione presentata a quest'Assemblea che impegna il Governo a concordare una strategia di azione con tutti gli operatori del settore ed a definire un sistema graduale di incentivi al fine di garantire una continuità di finanziamenti, in particolare, sul settore fotovoltaico. *(Applausi

aver consentito questo dibattito, peraltro anche su richiesta del nostro Gruppo parlamentare, e vorrei ringraziare il ministro Romani per essere presente. É chiaro che l'emendamento che il Governo ha presentato cambia la radicalmente politica energetica del Governo. Questa è una scelta che non può non essere oggetto di un dibattito pubblico, di un dibattito parlamentare, di un confronto sul merito delle questioni, perché è una scelta che comunque, nel breve, medio e lungo periodo, inciderà profondamente sul sistema economico produttivo del nostro Paese, sulla sua competitività a livello internazionale ed anche sulla politica estera del nostro Paese. Infatti dal punto

l'energia nucleare, dalla Francia, con cui com'è noto abbiamo ottimi rapporti, e dal resto dei Paesi che sono produttori di energia nucleare. Quindi, si tratta

convinto): «Oggi nessun Paese può rinunciare; non è possibile stare fuori alla possibilità di creazione dell'energia dell'atomo ed entro questa legislatura metteremo la prima pietra sulla prima centrale nucleare». Stesse dichiarazioni sono state rese dal suo predecessore, il ministro Scajola: «Il programma italiano per l'energia nucleare procede secondo la tabella di marcia e nel 2013 comincerà la costruzione della prima centrale. Il nostro programma nucleare è complesso, procede nei tempi previsti. Il Parlamento italiano ha approvato tutta la legislazione...». E vi risparmio il resto. Anzi, addirittura il Presidente del Consiglio, con la sua solita, ovvia e anche professionale dimestichezza con la comunicazione pubblica, ha proposto un progetto con la RAI per alcuni *spot* mirati a convincere gli italiani della sicurezza di nuove centrali nucleari che il Governo ha intenzione di costruire.

«Sono reduce», diceva entusiasta la Ministra «dagli incontri parigini per gli accordi sul nucleare e sono sempre più convinta. Si dovrebbero organizzare dei pellegrinaggi per andare a vedere come vivono le famiglie accanto agli impianti nucleari francesi. I territori che ospitano gli impianti hanno molte compensazioni: tasse, costo dell'energia», e anche la tinteggiatura verde; diceva così, insomma, di tutta la politica energetica anche del Governo francese, oltre che di quello italiano. le dichiarazioni rese dopo la tragedia di Fukushima: «Seguiamo con dolore», cito sempre testualmente il ministro Prestigiacomo «e preoccupazione le vicende giapponesi, ma trovo la polemica italiana offensivamente macabra. Gli impianti di Fukushima sono costruiti con una tecnologia vecchia di cinquant'anni, molto diversa dalle centrali di terza generazione che saranno costruite nel nostro Paese». In questo contesto, ancora, la ministra Prestigiacomo (Ministro dell'ambiente: lo ricordo per chi non lo sapesse) sosteneva: «La linea italiana rispetto al programma nucleare chiaramente non cambia. Seguiamo con sgomento la situazione in Giappone, senza nessuna sottovalutazione, ma neanche si deve speculare. Non era ancora finito l'effetto dello *tsunami* che già in Italia gli antinuclearisti sfruttavano

è cambiata radicalmente ed irreversibilmente la scelta del Governo che ha cancellato dal piano energetico nazionale il nucleare per ieri, oggi e domani. Infatti, dobbiamo stare agli atti e non alle interpretazioni: l'emendamento che voi avete presentato ricopia esattamente il quesito referendario e quindi abroga, da tutto il *corpus* legislativo in materia di energia, energia, il nucleare. All'esito della votazione che faremo nel pomeriggio in Parlamento, il nucleare sarà cancellato definitivamente, così come lo è stato all'esito del *referendum* del 1987 dal dibattito (perché noi non abbiamo centrali), dalla ricerca e dalle scelte di politica economica che noi anche abbiamo sostenuto per tentare di rendere più autonoma e quindi più sicura l'economia del nostro Paese e anche rendere meno costosa la produzione di energia, soprattutto per le famiglie italiane e per i cittadini italiani. questo, perché dobbiamo giocare a carte scoperte. La vostra decisione, che ha modificato il testo dell'articolo 5 che prevedeva una sospensione delle procedure di localizzazione e realizzazione degli impianti per un anno, la cosiddetta moratoria, moratoria, è stata presa non per paura - come lei in qualche modo ha voluto anche adombrare - del disastro nucleare di Fukushima, ma per paura del *referendum*. Allora è chiaro, ne prendiamo atto: voi avete paura del confronto elettorale, avete paura di un dibattito pubblico in cui ci si schieri su questi temi. Noi abbiamo un'idea, voi ne avete un'altra, l'avete cambiata. È lecito cambiare idea; non è lecito cambiare idea per convenienza e non per convinzione, e non è lecito non affrontare un dibattito dal punto di vista politico che sia trasparente e pubblico su temi che riguardano la vita e il futuro dei nostri figli e del nostro Paese. Proprio per questa ragione, signor Ministro, lei comprenderà che voi avete tentato di applicare - e non bene - una vecchia regola democristiana che diceva sostanzialmente questo: un problema rinviato è mezzo risolto.

ogni questione che si mette in mezzo al nostro cammino e che possa in qualche modo essere d'intralcio alla sopravvivenza di questo Governo; decidiamo di non decidere; bivacchiamo con la complicità di più o meno interessati e responsabili parlamentari del nostro Paese. La questione fondamentale è una: in questo Paese il problema più grave che abbiamo, come abbiamo scoperto a seguito dell'applicazione della regola di Scilipoti, è la legge sull'agopuntura. Allora occupiamoci, in questi due anni di legislatura, della medicina omeopatica e dell'agopuntura, tanto caldeggiata dal programma di governo di

del Paese; rifacciamoci una nostra piccola grande IRI con la Cassa depositi e prestiti, come stiamo facendo in questo decreto; anziché regolare il mercato, facciamoci noi il mercato, tanto abbiamo da tempo questa cultura, e chi presiede questo Governo più degli altri; godiamo quindi di questa spensierata insipienza, che porterà il vascello a navigare: fino a quando sul vascello ci siamo noi bene, poi il resto si vedrà. È un po' come la decisione

cioè l'abrogazione di norme che riguardano il nucleare, la cancellazione anche della ricerca, dell'approfondimento, della ricerca sulla ricerca, e quant'altro. Non mi riferisco alla realizzazione di centrali, anche se a sentire scienziati come Margherita Hack, che certamente è un'ambientalista, e non mi sembra sia una furiosa nuclearista, o altri, a cominciare dal professor Veronesi, dal professor Veronesi, appare impossibile che si possa verificare dal punto di vista geologico una tragedia come quella di Fukushima nel Mediterraneo. Certamente Fukushima pone un problema, perché tutti gli incidenti nucleari che ci sono stati al mondo fino ad ora sono stati frutto di un errore umano; per la prima volta siamo in presenza di un errore progettuale. L'errore progettuale è stato quello di sottovalutare il rischio del verificarsi di uno tsunami,

delle emozioni e mai sottoporre a strumentalizzazioni o a sciacallaggio politico» - come ha detto il Ministro dell'ambiente - «scelte che riguardano il futuro economico e sociale e delle imprese di questo Paese». Voi avete fatto l'esatto opposto: anziché porvi il problema di un approfondimento delle condizioni di sicurezza, ci consegnate a Sarkozy per l'energia atomica, alla Libia e alle sue tensioni, e a Putin per quanto riguarda l'approvvigionamento del gas. Tutto ciò avrà un impatto negativo sui conti del nostro Paese, sul bilancio delle famiglie, e questa è una bolletta che paghiamo grazie alla vostra azione e alla vostra inazione di Governo. Signora Presidente, la sicurezza è misurata in termini di rischio e il rischio dipende dalla sicurezza della macchina e dell'infrastruttura di sostegno e, quindi, dalla natura di affidabilità della stessa della stessa ed è misurabile con test da fatica e da stress che, se superati, rendono l'impianto sicuro. Ciò è capitato a Chernobyl dove il 26 aprile 1986, in seguito ad errori del personale, irresponsabilità dei dirigenti ed errori di progettazione, durante l'esecuzione di un test nella locale centrale elettronucleare, nel corso di una simulazione di guasto al sistema di raffreddamento, le barre di uranio del nocciolo del reattore nucleare si surriscaldarono per davvero fino alla fusione del nocciolo del reattore 4, con due conseguenti esplosioni. Una seconda sorgente di rischio naturale sono, ad esempio, terremoti e maremoti con conseguenti tsunami. il caso giapponese di Fukushima. È del tutto evidente che questo è un rischio più difficile da valutare. Infatti, nel caso specifico del Giappone, la centrale ha superato il rischio del terremoto, pur essendo il terzo per intensità misurato al mondo nella storia dell'uomo (magnitudo 9), ma non era stato previsto che l'onda dello tsunami, alta 14 metri, avrebbe messo fuori uso i contatti elettrici e le pompe per il sistema di raffreddamento dei reattori, provocando quindi il surriscaldamento delle barre di combustibile fino alla parziale fusione di alcune di esse. Ragionando pertanto con freddezza e lucidità, possiamo affermare che la tecnologia per la produzione di energia elettrica con l'atomo è sicura. Ringrazio il signor Ministro per le spiegazioni che ci ha fornito perché, alla luce di quanto ho appena finito di dire, se noi se noi affrontassimo questo dibattito con serenità credo che, valutate le ragioni di sicurezza, avremmo svuotato il dibattito. In realtà, non è così, perché la scelta sul nucleare, come è stato detto e scritto, come pure la presentazione dell'emendamento 5.800, non sono motivate da ragioni scientifiche, ma da opportunità politiche. È evidente che un *referendum* in queste condizioni di emotività, non solo per il disastro di Fukushima ma anche per il modo in cui si affrontano da anni questi temi in Italia, avrebbe segnato definitivamente l'uscita dell'Italia da questo tipo di tecnologia. Non mi riferisco alla costruzione degli impianti, ma allo sviluppo della ricerca. Il modo politico dissennato con cui noi ci avviciniamo al *referendum*, peraltro, è testimoniato da una serie di *e-mail* che sono arrivate alla nostra posta elettronica in questi giorni, nelle passate settimane.

rispetto a ciò che è stato detto fino ad oggi, ma è l'unico modo che noi abbiamo di salvare la ricerca in questo settore. Io spero che in futuro possano svilupparsi centrali nucleari in Italia), perché, se passasse il *referendum*, ci troveremmo esattamente nella situazione in cui, unico Paese al mondo, ci siamo trovati negli anni passati. negli Stati Uniti non hanno pensato di non costruire più centrali nucleari. Dopo Chernobyl, nel resto del mondo, non si è pensato di non costruire più centrali nucleari,

il *referendum* del prossimo giugno, rischieremmo di trovarci nella stessa situazione. Quindi, secondo me, bene ha fatto il Governo a proporre questo emendamento

con un nuovo piano energetico, potremo finalmente dare risposte ai bisogni energetici dell'Italia anche attraverso l'introduzione del sistema di produzione di energia elettrica attraverso l'atomo.

in cui verrà distribuito ai senatori il bilancio interno del Senato.

per una trasfusione errata di plasma, è una di quelle oltre 7.000 persone che avevamo chiesto di attenzionare, di rispettare

domande per vedere rivisti i loro diritti agli indennizzi. In questa articolata interrogazione avevamo suggerito cose importanti al Ministero e avevamo chiesto di sapere come stanno andando le nuove pratiche e i nuovi indennizzi. L'interrogazione era del giugno 2010; chiediamo adesso con molta urgenza e determinazione che questa risposta ci sia data,

volte a considerare il comportamento dei parlamentari come macchiettistico - e non dico altro - si legge anche: «La passione per la tavoletta è trasversale: tutti i deputati e i senatori di qualunque partito lo hanno avuto in dono lo scorso Natale dai rispettivi partiti, pagato con i soldi degli italiani (il modello base costa circa 500 euro)».